saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Marisa Salerno in Masciari, Francesco e Ottavia sono una famiglia calabrese sottoposta a programma di protezione in quanto Pino è testimone di giustizia dal 1996, dopo che da imprenditore ha denunciato il ricatto estorsivo della criminalità organizzata, diventando testimone dei principali processi contro la 'ndrangheta e facendone condannare i *boss*, nonché gli esponenti politici e della magistratura collusi al sistema estorsivo. Pino Masciari è invitato a parlare di giustizia e legalità in diverse località d'Italia da scuole, associazioni, istituzioni locali, venendo riconosciuto l'alto valore della sua esperienza, avvalorato dalla limpidezza dimostrata nelle sue testimonianze processuali come riconosciuto in diverse occasioni ufficiali. La sua storia di imprenditore onesto e abile (e il notevole fatturato ne era dimostrazione) che denuncia tutto un apparato marcio facendo nomi e cognomi dei singoli e smontando, quindi, un intero sistema, è arrivata al punto da far condannare, perché partecipe all'estorsione, un consigliere di Stato, Saverio Damiani, poi interdetto dai pubblici uffici. La stessa delibera della commissione «Masciari, imprenditore edile, ha reso un eccezionale contributo testimoniale all'autorità giudiziaria consentendo la disarticolazione delle pericolose organizzazioni criminali che si erano rese responsabili di continue estorsioni e vessazioni ai suoi danni con estremo coraggio, rompendo un muro di tradizionale e di impenetrabile omertà, ha reso decisive dichiarazioni accusatorie a carico dei soggetti responsabili, tra i quali anche pubblici amministratori che avevano imposto tangenti sugli appalti, i quali sono stati condannati proprio sulla base delle sue dichiarazioni Evidenziata l'importanza e la rilevanza del contributo offerto dal predetto all'autorità giudiziaria, per la particolarità del contesto nel quale si inserisce e per il coraggio dimostrato, tale da aver assunto indiscusso risalto ed un valore simbolico, come riportato da altri organi istituzionali,

il coraggio della scelta testimoniale e l'alto prezzo personale pagato in conseguenza di ciò riconoscono l'unicità del caso quale primo atto concreto di fare antimafia: il cittadino onesto al servizio dello Stato. Pino Masciari è nota perché è stata discussa più volte. Persiste però l'assenza di un protocollo di sicurezza e di tutela indirizzato al caso, costante e non precario, a singhiozzi, come sta avvenendo.

che: «ci sono negozi in centro a Firenze che chiudono, perché la richiesta di pizzo supera il canone mensile d'affitto». Nel verbale di comunicazione, riportante il contenuto della nota n. 70714, in cui la commissione centrale comunica che le «istanze presentate, con le quali ha chiesto l'accompagnamento e scorta durante i suoi viaggi, (...) che avranno luogo nel periodo 19 settembre - 19 ottobre 2008, non sono state accolte. Il teste potrà, in ogni caso, effettuare tali spostamenti in piena autonomia». E con pericolo alla sua sicurezza. Le contraddizioni di ciò si riassumono nella delibera del 2 ottobre 2008 che recita: «il testimone di giustizia Masciari Giuseppe, fino alla definizione del giudizio amministrativo riguardante l'impugnativa della delibera di fuoriuscita dal programma, è a tutti gli effetti inserito nel programma speciale di protezione e, in relazione a tale condizione, ha il dovere di collaborare con le autorità preposte alla sua sicurezza, per evitare ogni ipotetico rischio derivante dal suo *status*»; egli ha impugnato la delibera del 27 ottobre 2004 proprio perché non erano previste misure di sicurezza, esponendo lui e la sua famiglia a rischio di vita, che non è venuto meno. La commissione aveva escluso già da allora ogni forma di protezione con l'esclusione dal programma di protezione, ribadendo tale concetto nella richiamata delibera dell'1 febbraio 2005, che rimarca ancora una volta che, alla mancata accettazione della delibera del del soggetto, seguirà comunque una cessazione del programma speciale di protezione. La delibera del 2 ottobre 2008 cita: «Il Masciari sarà comunque sottoposto a un dispositivo di sicurezza a cura del servizio centrale di protezione». Non specifica dunque quali sono i dispositivi da predisporre in merito alla sua sicurezza, evidenziando così un atteggiamento di mera giustificazione per sé, ma non di reale interessamento alle condizioni di esposizione al rischio, in quanto il termine «dispositivo di sicurezza» risulta generico. Mi avvio alla conclusione, signora Presidente. Agli appuntamenti di San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo, Roma, Torino, Santa Margherita in Belice e Bologna, si è verificata l'assenza completa di tutela e scorta. Agli appuntamenti di Udine c'è stata una presenza di forze dell'ordine; a Catanzaro c'è stata scorta di tutela. A Torino, il 10 novembre, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria, Pino Masciari è stato raggiunto da 5 agenti competenti con due vetture adeguate, situazione poi svilita dall'arrivo di un unico mezzo obsoleto e insensato per spostare una famiglia di 4 persone e 2 agenti; solo *in extremis* per la presenza di vetture civili. Insomma, non c'è coerenza nelle decisioni riguardanti la sicurezza di Giuseppe Masciari e della sua famiglia.

dei cittadini, a maggior ragione dei soggetti già sottoposti a programma di protezione, che risultano in evidente rischio di vita. Infine di prendere in considerazione la possibilità di nominare Giuseppe Masciari *testimonial* di legalità e giustizia, figura ufficiale prevista dalla legge n. 45 del 2001, come già effettuato in altri casi e per altri soggetti da lui stesso nominati. PRESIDENTE. Il rappresentante

Uno dei limiti principali della legge n. 91 del 1992, che fino al 2001 aveva disciplinato il sistema delle protezioni, è stato quello della mancata distinzione tra i collaboratori di giustizia - i cosiddetti pentiti e i testimoni, ovvero tra chi, al di là dei drammi interiori, ha commesso delitti e punta ai premi derivanti dalla collaborazione e chi, persona onesta, non può e non deve subire danni per le dichiarazioni che rende su gravi fatti criminali. Il risultato è stato che per troppo tempo - circa un decennio - i testimoni di giustizia sono stati considerati alla stregua dei cosiddetti pentiti, con profonde ferite della dignità personale, unitamente a gravi disfunzioni operative. Ritengo di aver avuto una minuscola parte nella modifica di questo sistema: ho infatti redatto nel corso della XIII legislatura, per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, una relazione sui testimoni di giustizia, approvata all'unanimità nel 1998, nella quale si descrivevano queste anomalie, partendo dall'esame di casi concreti. Ho inoltre presentato, sempre nel corso della XIII legislatura, una proposta di legge tesa al riconoscimento di un vero e proprio statuto del testimone di giustizia: esso è stato recepito nella legge n. 45 del 2001 di riforma del sistema di protezione. Quella legge ha introdotto profonde innovazioni in materia, partendo dal presupposto che i testimoni di giustizia non hanno soltanto un indubbio valore processuale, dal momento che la loro parola non necessita a stretto rigore di riscontri, ma hanno un valore civile ancora più certo, soprattutto nelle aree di consolidata tradizione omertosa, nelle quali sono rari i casi di testimoni oculari di delitti. Proprio per questo, la legge di riforma ha differenziato in modo netto la posizione dei testimoni da quella dei collaboratori, con disposizioni a tutti note. La legge, poi, è stata seguita nel 2004 da un decreto ministeriale costituente regolamento di attuazione. Dall'ottobre del 2001 fino al maggio 2006, e poi nuovamente a partire dal luglio di quest'anno, sono stato e sono chiamato quotidianamente ad applicare queste norme quale presidente della commissione sui programmi di protezione. Nel periodo intermedio, tale compito è stato svolto dall'onorevole Minniti, quale vice ministro dell'interno. Voglio ricordare questo per sottolineare l'assoluta continuità: non si parla di questo o di quel Governo, si parla dello Stato e della sua posizione nei confronti dei testimoni di giustizia. In tale veste posso dire con assoluta serenità - ma cercherò di documentarlo con qualche dato - che negli atti di sindacato ispettivo vi è una serie di inesattezze. Dall'insieme di norme primarie e secondarie varate a seguito della legge del 2001, i testimoni di giustizia non hanno un trattamento parificato o addirittura inferiore a quello dei collaboratori di giustizia. Ci sono, com'è ovvio che sia, delle differenze importanti positive. I testimoni di giustizia, per esempio, hanno accesso a mutui agevolati senza dover prestare garanzie, in virtù di una convenzione stipulata con un importante istituto bancario, e ciò non accade per i collaboratori; hanno facoltà di chiedere allo Stato l'acquisizione, a prezzo di mercato, dei beni che lasciano nella località d'origine, se sono trasferiti, e anche questo non accade per i collaboratori; possono inoltre servirsi di consulenti di loro fiducia, le cui prestazioni sono interamente a carico del Servizio centrale di protezione, per qualsiasi problema legato alle pregresse attività di lavoro e a quelle future da intraprendere; ricevono assegni mensili di mantenimento di importo superiore del 50 per cento - sulla base di criteri oggettivi contenuti in una delibera della commissione - a parità di consistenza del nucleo familiare, rispetto ai collaboratori di giustizia, con possibilità di integrazioni maggiori in presenza di un reddito pregresso documentato. Godono del rimborso delle cure mediche, comprese quelle odontoiatriche, effettuate in regime privatistico, di contributi straordinari relativi al tenore di vita preesistente (rimborso vacanze, acquisto testi e attrezzature scolastiche) e della possibilità - com'è giusto che sia - di visionare preventivamente gli alloggi scelti per loro dal Servizio centrale di protezione, che sono sempre di livello almeno pari a quello occupato nella località d'origine. Possono inoltre fruire, a richiesta, di colloqui di orientamento e di sostegno con i direttori tecnici psicologi del Servizio centrale di protezione, e del risarcimento del danno biologico, in merito all'accertamento del quale vige da tempo una convenzione col servizio medico-legale dell'INPS. Dall'approvazione della legge n. 45 del 2001 si è molto lavorato sul terreno del reinserimento socio-lavorativo del testimone, nella consapevolezza che esso non può prescindere, così come prescrive la legge, dal tenore di vita e dal tipo di attività che ha preceduto l'ingresso nel programma di protezione. Il discorso è relativamente più agevole quando il testimone in precedenza ha svolto un lavoro autonomo (per esempio ha gestito un esercizio commerciale o ha condotto un'azienda), mentre presenta aspetti più problematici nell'ipotesi in cui l'attività antecedente alla deposizione era alle dipendenze dei privati; ma anche da questo punto di vista si è lavorato per reinserire chi aveva questa condizione pregressa. La trattazione dei singoli casi riguardanti i testimoni è avvenuta e avviene col coinvolgimento attivo degli stessi interessati, ai quali è chiarito nel corso delle audizioni svolte in commissione, che non devono in alcun modo sentirsi controparte rispetto allo Stato, bensì protagonisti delle scelte relative al proprio futuro, contribuendo in modo propositivo alla formazione della decisione che li riguarda. Le audizioni, peraltro, permettono alla commissione di avere l'esatta cognizione della condizione dei testimone di giustizia e quindi di poter adottare i provvedimenti ritenuti più aderenti alla soluzione dei problemi rappresentati. Sui testimoni giochiamo una partita difficile: quella della credibilità delle istituzioni nella lotta alla criminalità. La garanzia di un adeguato futuro ai testimoni e alle loro famiglie è in grado di incoraggiare altri a non avere remore nel riferire quanto è a propria conoscenza alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria. Obiettivo primario, peraltro, è consentire il più possibile, se ovviamente il testimone lo desidera o lo chiede, la permanenza nel luogo di origine attraverso misure adeguate delle quali, in ogni caso, va sempre verificata la possibilità.

Questa, a mio avviso, è una vittoria dello Stato pur nelle obiettive difficoltà di tutela, perché quando un testimone viene ammesso al programma, la sua protezione, con trasferimento in una località protetta è garantita Si porta il testimone a 1.000 chilometri di distanza in un luogo dove nessuno, perlomeno in teoria, lo conosce. La protezione *in* *loco*, dove invece è conosciuto, richiede un meccanismo di tutela imponente per uomini

di garantire il minor disagio possibile al testimone, ma anche di trasmettere un messaggio di forte presenza dello Stato, che non costringe chi collabora per l'accertamento dei fatti delittuosi ad allontanarsi e a lasciare il luogo d'origine. Intendo, più in generale, ricordare un solo dato relativo all'applicazione della nuova legge. Si tratta del dato riguardante le nuove ammissioni ai programmi di testimoni di giustizia dal momento in cui è iniziata l'applicazione della legge n. Nel periodo compreso tra il secondo semestre 1996 e il primo semestre 2001, quindi prima che entrasse in vigore la legge, i nuovi testimoni ammessi al programma furono complessivamente 27, in media poco più di cinque all'anno. Dalsecondo semestre 2001, ossia da quando è operativa la nuova legge fino ad oggi, le nuove ammissioni sono state 116, con una media di più di sedici all'anno e cioè più del triplo rispetto a prima del varo della legge n. 45 del 2001, a dimostrazione del successo delle nuove disposizioni.

viene ammesso al programma di protezione, con delibera della commissione centrale, il 17 marzo 1998, su proposta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Nel programma erano inclusi la moglie e i due figli minori, che non cito per nome. L'imprenditore aveva riferito, in qualità di testimone, di essere stato oggetto di estorsioni che gli avevano provocato una grave esposizione debitoria, anche per effetto dei prestiti usurari contratti nei confronti di appartenenti ad organizzazioni criminali, ai quali era stato costretto a rivolgersi. Tale situazione debitoria aveva provocato il dissesto della sua impresa e quindi la dichiarazione di fallimento nell'ottobre del 1996. Non risponde al vero che è mancato il sostegno per l'inserimento lavorativo della moglie di Masciari, odontoiatra. La signora, infatti, ha ricevuto, poco dopo l'ingresso nel programma, un contributo pari a lire (all'epoca vi erano le lire) 388.631.000, oltre alle spese necessarie per il trasferimento delle attrezzature di lavoro. Tale contributo è stato incassato e mai utilizzato secondo la destinazione, nonostante la legge preveda che esso debba essere impiegato e che l'impiego debba essere documentato. Ella ha, altresì, rifiutato di lavorare presso una ASL, lavoro che le era stato procurato, ed ha altresì rifiutato un impiego in uno studio privato e una collaborazione di odontoiatra con un docente universitario. Non risponde al vero che è mancato il sostegno per il reinserimento lavorativo di Masciari. È vero il contrario. Proprio al fine di permettere il pieno reinserimento nella vita economica e sociale, la commissione ha anzitutto acquisito elementi che provassero il collegamento tra l'estorsione e l'usura subita e il precipitare della sua condizione fino al fallimento. Tali elementi in origine erano assenti. Inoltre, ha puntato ad articolare una via d'uscita al fallimento, in assenza della quale il pregiudizio a suo danno derivante dalle inibizioni collegate allo *status* di fallito avrebbe precluso ogni seria ripresa di attività. Ciò ha impegnato la commissione in un lungo e complesso lavoro di audizioni e di contatti fra i vari soggetti istituzionali interessati, colmando lacune comunicative da parte di più di un ufficio giudiziario e colmando documentazioni inadeguate da parte di Masciari. Fra il 2001 e il 2004 la commissione ha ascoltato in audizione Masciari per ben sette volte (per brevità evito di citare le date). La commissione ha, altresì, ascoltato in audizione il giudice delegato e il curatore del fallimento di Masciari il 22 gennaio 2003. Il 6 ottobre 2004 ha ascoltato, sempre in audizione, il pubblico ministero delegato a seguire i procedimenti che interessavano Masciari quale testimone. Benché il magistrato avesse sostenuto che il collegamento fra la testimonianza e il fallimento non fosse munito di specifici riscontri, tuttavia la circostanza che alcuni immobili, già intestati alla Masciari Costruzioni, fossero nella disponibilità degli imputati da lui accusati ha fatto propendere autonomamente la commissione per una indiretta conferma del nesso causale tra le estorsioni subite e l'esposizione debitoria che aveva condotto al fallimento. Tale conclusione, lo ripeto, è stata frutto di un approfondimento svolto dalla commissione, non dall'autorità giudiziaria proponente. A seguito dell'istruttoria complessa prima descritta, il 27 ottobre 2004 a Masciari è stata proposta una definizione della posizione nei termini che seguono: il Servizio centrale di protezione è stato incaricato di porre a disposizione degli organi del fallimento

di erogare a Masciari, a chiusura (cioè dopo la procedura concorsuale e non prima, altrimenti ci sarebbe stato l'assorbimento dal passivo fallimentare) della capitalizzazione delle misure di assistenza economica nella misura massima prevista dalle determinazioni riguardanti i testimoni di giustizia. In base al decreto ministeriale la capitalizzazione può avvenire da un minimo di due anni di assegno mensile di mantenimento (con tutte le integrazioni, locazioni eccetera) fino ad un massimo di dieci anni. Per Masciari è stata proposta la misura massima di dieci anni per un totale di 267.400 altresì incaricato di erogare a Masciari e alla moglie, a chiusura della procedura concorsuale, le somme determinate a titolo di danno biologico risultanti dalla perizia medico-legale dell'INPS, eseguita su incarico della commissione, sulla base delle tabelle del tribunale di Roma secondo gli indici ISTAT, pari rispettivamente a euro 18.870 euro per Masciari e a 29.670 euro per la moglie; moglie; di fare salvi gli effetti della delibera del 23 marzo 2000, in quanto finalizzata alla realizzazione del reinserimento sociale della moglie di Masciari, e quindi di mantenere a suo favore il contributo straordinario all'epoca erogato di 388.631.000 lire, oltre a quelli necessari per il trasporto e il montaggio delle attrezzature; di prorogare, nelle more della definizione della procedura concorsuale, il programma speciale di protezione nei confronti di Masciari e del suo nucleo familiare per ulteriori cinque anni a decorrere dal marzo 2000 (siamo all'ottobre del 2004), fatte salve nuove determinazioni. La commissione non si pronunciava sul mancato guadagno di cui all'articolo 16-*ter* della legge sui collaboratori di giustizia, ritenendo gli elementi informativi acquisiti, in assenza di un valido contributo da parte dell'interessato, insufficienti per pervenire alla valutazione; l'accertamento, però, limitatamente a tale aspetto, veniva demandato al commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, organo competente in merito alla concessione delle provvidenze relative. Quindi, non vi era un rifiuto a considerare tale aspetto (il mancato guadagno), ma un rinvio all'autorità competente, peraltro più volte presente in commissione per esaminare congiuntamente alla commissione il caso e, quindi, a conoscenza dello stesso anche nel dettaglio. Contro questo provvedimento Masciari e la moglie hanno presentato ricorso al TAR del Lazio ed il TAR del Lazio fino ad oggi non si è pronunciato. credo vada sottolineato - non ha causato nessun danno a Masciari, il quale è rimasto nella pienezza del programma di assistenza e protezione, in attesa della definizione del giudizio. Concludendo sul punto, il reinserimento di Masciari sarebbe avvenuto già più di quattro anni fa se lo stesso Masciari non avesse rifiutato, impugnandola, la delibera della commissione che riportava le voci prima elencate; e sarebbe avvenuto restando impregiudicata la protezione personale e la definizione del mancato guadagno, per un importo complessivo di 1.810.069,76 euro. Lo Stato, quindi, già quattro anni fa, ha proposto a Masciari, ricevendo un rifiuto, una definizione non inferiore a 1.800.000 euro. La sua posizione è stata ripresa sotto il precedente Governo dalla commissione presieduta dal Vice ministro, onorevole Marco Minniti. Essa ha nuovamente disposto, il 29 novembre 2006, l'audizione di Masciari alla presenza della moglie e dei legali. In quella sede, l'interessato ed i legali insistevano per l'individuazione della voce «mancato guadagno» anche a titolo transattivo, in pendenza del ricorso al TAR e chiedevano, a tal fine, la costituzione di un tavolo tecnico per elaborare i relativi parametri di valutazione. Il tavolo tecnico veniva istituito e nel corso dei suoi lavori - tenutisi il 17 e il 31 gennaio 2007 e l'11 giugno 2007 - veniva individuato quale possibile parametro di riferimento per l'accertamento del mancato guadagno il valore medio del volume di affari dell'impresa del testimone di giustizia, risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalla documentazione relativa alla sentenza di fallimento del tribunale di Vibo Valentia, quale indicatore obiettivo per ricostruire le possibilità di sviluppo e la conseguente redditività dell'impresa del testimone, facendo ricorso a studi specifici nel settore dell'edilizia. Né Masciari, né i suoi legali, benché sollecitati, hanno mai fatto conoscere le proprie indicazioni o documentazioni in ordine a quanto prospettato nel corso delle riunioni del tavolo tecnico. Masciari nel luglio del 2007 ha presentato un progetto di reinserimento lavorativo che riteneva confacente alle esigenze proprie e della famiglia, relativo alla proposta di acquisto di una struttura alberghiera del costo di circa 4,5 milioni di euro, più oneri fiscali. In ragione dell'entità dell'investimento e della complessità dell'operazione economica, la commissione disponeva, con delibera del 17 dicembre 2007, di incaricare un professionista al fine di verificare la stima e la congruità del valore del compendio immobiliare oggetto della proposta di acquisto. È stato, altresì, dato incarico al consulente della commissione ed al segretario di essa di svolgere attività di raccordo al fine di accelerare l'attività istruttoria. Sono stati svolti anche dei sopralluoghi. Dalla relazione compilata dal professionista emergeva con estrema chiarezza una valutazione negativa dell'attività in questione. alla luce dei bilanci definitivi disponibili nel triennio 2004-2006, la società cedente questo albergo risultava aver costantemente realizzato non utili, bensì perdite di esercizio e non vi erano elementi oggettivi per stimare la realizzazione di un potenziale reddito prospettico, anche nel caso in cui l'acquisto fosse avvenuto al netto di oneri finanziari, che però gravavano sull'azienda. Qualora poi si fosse inteso prendere a riferimento il risultato positivo dell'ultimo esercizio, pari a circa 60.000 euro, il reddito prospettico sarebbe stato comunque inferiore al capitale investito nell'impresa e, pertanto, non remunerativo. Inoltre, da parte dello stesso cedente dell'albergo si stava profilando un'iniziativa imprenditoriale concorrenziale a breve distanza e meglio collegata con i servizi di pubblica utilità. Vogliamo chiamarlo un tentativo di truffa? Quindi, il rifiuto del progetto era nell'interesse dello stesso Masciari, che non avrebbe potuto far fronte alla gestione di un cespite anche potenzialmente, non solo attualmente, in passivo. Con delibera del 24 aprile 2008 la commissione confermava le valutazioni della precedente delibera dell'ottobre 2004 e incaricava il Servizio centrale di protezione di porre nuovamente a disposizione degli organi del fallimento 1.293.418,60 euro per la definizione del fallimento. Inoltre, erano previsti: per capitalizzazione 287.200 euro (la differenza rispetto a quella della precedente commissione è semplicemente l'indicizzazione ISTAT); per danno biologico grosso modo le stesse cifre (25.287 euro per Masciari 39.760 euro per la moglie); per mancato guadagno della moglie 200.000 euro abbondanti. Inoltre, erano previsti una somma forfetaria per i figli (200.000 euro), calcolata in via equitativa al ristoro dei disagi e di ogni altro danno, nonché il mancato guadagno (non soccorrevano i dati che si rinvengono nelle dichiarazioni dei redditi di Masciari in quanto evidenzianti utili netti modestissimi o inesistenti). Sulla base dei dati acquisiti e della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, si è determinata la redditività media dell'impresa - come si diceva prima - con caratteristiche analoghe nel settore e in base ad un complesso sistema di calcolo fondato su criteri di equità. A titolo risarcitorio si è pervenuti ad una quantificazione di mancato guadagno pari a 1.639.131,88 euro, con l'autorizzazione per Masciari e la moglie, previa loro richiesta, di avvalersi della convenzione per l'accesso a mutui a tassi agevolati per l'importo massimo di 300.000 euro, lasciando impregiudicato il diritto degli interessati a ottenere l'acquisizione di eventuali beni immobili di loro proprietà al patrimonio dello Stato e con la prosecuzione delle misure di protezione e di assistenza per un ulteriore biennio. Le misure di protezione erano assicurate anche per gli ulteriori impegni giudiziari cui Masciari dovesse essere chiamato insieme ad esse veniva confermata l'assistenza legale nei procedimenti nei quali sia eventualmente ancora chiamato a rendere dichiarazioni ovvero eserciti le facoltà e i diritti riconosciuti dalla legge quale persona offesa o parte civile. L'interessato e la moglie, all'atto della notifica di questa delibera, hanno apposto la dicitura «firmo per ricevuta della notifica con ogni più ampia riserva di azione». Il precedente presidente della commissione, preso atto di quanto sopra, ha comunicato al Servizio centrale di protezione che la delibera del 24 aprile 2008 risultava eseguibile solo con la piena e incondizionata accettazione da parte dell'interessato, previo il verificarsi delle condizioni in essa contenute. Contro la seconda delibera di capitalizzazione è stato presentato ricorso per motivi aggiunti con richiamo al ricorso pendente. Risulta fissata per il 18 dicembre 2008 l'udienza dinanzi al TAR del Lazio per la discussione del ricorso amministrativo proposto da Masciari e dalla moglie.

in presenza dell'ipotesi di definizione più ampia mai riconosciuta ad un testimone di giustizia: siamo in totale a 3.685.508,64 euro. La commissione, cioè lo Stato, ha posto a disposizione di Masciari più di tre milioni e mezzo di euro. Ripeto, la cifra più alta in assoluto mai proposta ad un testimone di giustizia. Masciari ha rifiutato. ha rifiutato. Da ultimo, non risponde al vero che Masciari sia rimasto privo di tutela. Intanto, ribadisco che in questo momento, in pendenza del giudizio amministrativo e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 10 della legge del 1991, così come modificata, il testimone è tuttora inserito nel programma speciale di protezione e, quindi, continua a fruire dell'assegno di mantenimento, dell'alloggio protetto e delle altre misure di assistenza e tutela previste per le persone soggette a programma speciale di protezione. Vorrei poi richiamare la delibera di massima sulle trasferte dei testimoni di giustizia adottata il 18 dicembre 2006 dalla precedente commissione, che quella attuale condivide (perché - lo ripeto - non stiamo facendo questione di Governi, ma di interlocuzione che avviene sempre con lo Stato), all'insegna della trasparenza e della conoscibilità. Con tale delibera la commissione ha disposto di inserire nel programma di protezione dei testimoni di giustizia, tra le misure di assistenza, una voce riguardante le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di pernottamento e di vitto (fatta eccezione per le spese extra, che restano a carico del testimone di giustizia) sostenute sul territorio nazionale: incondizionatamente, nel caso di trasferta per motivi di giustizia connessa alla testimonianza prestata, ivi compresi gli incontri con gli avvocati; sempre, nel caso di trasferta in località di origine, a condizione che sia stata previamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, che sia circoscritta sotto il profilo temporale e che non abbia carattere di periodicità, ciò per evidenti esigenze di sicurezza; solo a seguito di specifica autorizzazione della commissione, nel caso di trasferte per altri motivi. Sono state disciplinate anche le spese connesse alle ferie, di volta in volta valutate dalla commissione centrale anche alla luce del precedente tenore di vita del testimone e della congruità della somma richiesta, e che in ogni caso non superino il doppio dell'assegno di mantenimento. È stato stabilito che le spese sostenute dal testimone di giustizia a titolo diverso restino a carico esclusivo dell'interessato. Alla stregua di tale deliberazione, che risponde al criterio generale di correttezza nell'uso delle risorse pubbliche, cui tutti siamo tenuti, sono state decise negativamente di recente numerose istanze con le quali il Masciari e la moglie nel comunicare impegni in una località italiana e all'estero, a New York, per il *Columbus day*, hanno chiesto la corresponsione di somme in denaro trattandosi di impegni in località diversa da quella di origine per ragioni diverse da quelle di giustizia o da quelle strettamente familiari. La commissione ha quindi disposto che, qualora Masciari ritenga comunque di muoversi sul territorio nazionale, pur in contrasto con le cautele che sottendono all'esecuzione di ogni programma speciale di protezione, il medesimo continuerà a fruire di un dispositivo di sicurezza a cura del Servizio centrale di protezione; avrà quindi tutela senza alcun limite. E la tutela non è una cosa generica: è qualcosa che ha un contenuto specifico e significa protezione con uomini in macchine particolari. A carico del medesimo Servizio non graverà, invece, alcun altro onere (rimborsi, alberghi o altro) derivante da appuntamenti che non siano connessi ad eventuali impegni di giustizia del testimone, così come risulta dalla delibera prima ricordata. Non è da escludere che, come gli interroganti segnalano, Masciari in qualche circostanza si sia presentato privo di protezione, ma se ciò è accaduto protezione, ma se ciò è accaduto - non lo so - è avvenuto per una scelta deliberata e, se mi permettete, incauta dello stesso Masciari che, come tutte le persone sottoposte a tutela, è tenuto a comunicare i propri spostamenti a chi è preposto alla sua tutela. Lo sa molto bene il senatore Lumia che credo abbia avuto (non so se ne fruisca ancora) un dispositivo di tutela; lo sa chi sta parlando in questo momento e lo sanno tante altre persone, purtroppo. È una delle condizioni per le quali il meccanismo di tutela funziona. Spiace, infine, che, a seguito di queste polemiche che ruotano soprattutto attorno a Masciari e non alle altre decine di testimoni di giustizia, si veicoli l'immagine che, da un lato, vede presunti difensori del testimone di giustizia e, dall'altro, lo Stato che si mostrerebbe indifferente, se non ostile. Non vi sono fronti contrapposti, ma un unico e comune terreno di lotta contro la criminalità che vede la valorizzazione nei fatti - come dimostrano i dati - della figura del testimone di giustizia. Mi chiedo e chiedo agli interroganti, in spirito di costruttivo confronto, perché, a distanza di sette anni dall'approvazione di una legge che ha dato buona prova di sé (se è vero che le nuove ammissioni di testimoni sono più che triplicate), non si debbano valorizzare le positive esperienze di decine e decine di testimoni di giustizia pienamente inseriti che rappresentano la regola e che nel corso del programma non hanno avuto nulla da ridire sul comportamento della commissione, del Servizio di protezione e, quindi, dello Stato, nonostante la drammaticità della loro condizione. Resta fermo che l'intera attività della commissione sui programmi di protezione può essere in qualsiasi momento esaminata dal Parlamento, come è già avvenuto in più occasioni ad opera della Commissione parlamentare antimafia, la cui procedura è più che idonea a garantire questo tipo di interlocuzione perché svolge audizioni non pubbliche e, quindi, permette anche di ostendere dati riservati, mentre le informazioni sull'intero sistema sono fornite semestralmente al Parlamento dalla relazione che per legge il Servizio centrale di protezione trasmette alle due Camere.

già affrontato alla Camera, è bene ritornarci anche qui al Senato perché il tema che trattiamo è molto delicato; è un tema difficile e complesso, una sfida seria per lo Stato. ha richiamato più volte, sia alla Camera sia oggi pomeriggio al Senato, la necessità di sentirci Stato in continuità, al di là dei Governi che si succedono alla guida del Paese, e anche di sentirci Stato unitario, al di là delle appartenenze che fanno parte della vita ordinaria della politica democratica italiana. Condivido pienamente questo approccio, questo approccio, che però non si svolge secondo l'idea che ha riproposto anche qui stasera il sottosegretario Mantovano. Non c'è nessun allarme strumentale, non c'è nessun atteggiamento negativo; c'è semmai un giudizio critico preoccupato, leale e documentato. Lo Stato, in continuità e unitariamente, ha rilevato più volte che sui testimoni di giustizia si è agito male, con sufficienza e con errori. Abbiamo una vasta documentazione a tale proposito: è la storia della Commissione parlamentare antimafia recente che lo testimonia.

In quella relazione, onorevole Mantovano, lei stesso faceva riferimento alla condizione preoccupante

che oggettivamente scoraggiano ipotesi di collaborazione, mettere mano ad una nuova legge». Ecco perché non c'è nessun atteggiamento strumentale, nessun allarme. Lei stesso ne ha parlato nella Commissione parlamentare antimafia, con una relazione che fu approvata all'unanimità.

e soprattutto la parte riferita ai testimoni trovò un'amplissima convergenza. Si tratta di un risultato positivo, di una buona legge, spesso però applicata male, tant'è vero che la Commissione parlamentare antimafia è dovuta ritornare sempre sui testimoni di giustizia. L'apposito Comitato della XIV legislatura

anche in quell'occasione furono espresse valutazioni preoccupate e critiche sulla gestione dei testimoni di giustizia. In quella relazione si ricorda che ci sono due visioni differenti. Si usa questo linguaggio: «Nel documento vengono evidenziate le differenze che emergono dal raffronto tra la documentazione prodotta dal testimone audito e quella consegnata dal Servizio centrale di protezione. Con ogni probabilità, si afferma nel documento, tali differenze costituiscono espressione di due diversi modi di percepire la medesima situazione e dunque espressione di due diverse sensibilità alle problematiche che affliggono la vita di chi decide di rendere testimonianza dei fatti di cui è a conoscenza, spesso per essere per essere stato vittima inconsapevole». E si cita proprio il caso Masciari: «Giuseppe Masciari. Relazione all'esito della documentazione presentata nel corso di un'audizione l'11 novembre 2004». Ma non finisce qui. Visto che la condizione dei testimoni, non solo relativamente al caso Masciari, ma a diversi altri, è emersa in tutta la sua drammatica evidenza

Anche in quel contesto ci siamo espressi in modo unitario, Governo di centrosinistra e relazione firmata da una deputata dell'opposizione, l'onorevole Angela Napoli. Anche in quell'occasione, Presidente, si sono espressi giudizi molto severi e documentati sulla condizione dei testimoni di giustizia. Si fa riferimento alla scarsa assistenza, specie nella fase iniziale di ammissione alla speciale protezione, a chi abbandona un modo di vivere per assumerne un altro completamento diverso. Si fa riferimento a situazioni familiari talvolta complesse che non hanno trovato opportuna assistenza. Si fa riferimento alla limitata capacità degli organi di protezione a trattare testimoni che svolgono l'attività di imprenditorie nella località di origine e avrebbero voluto continuare a svolgerla anche nella realtà protetta. Ancora, si fa riferimento alle difficoltà a cambiare generalità, anche quando la situazione autenticamente lo richieda. Si fa riferimento a capitalizzazioni anticipate, che sembrano aver perso la loro reale finalità, connessa a un effettivo recupero del testimone nell'ambito lavorativo e sociale. Si fa riferimento a minacciata sicurezza nei luoghi protetti, in quanto i testimoni di giustizia mantengono, anche per esigenze connesse al pregresso mondo del lavoro, dipendendo da situazioni patrimoniali familiari con strascichi e con altre condizioni che permangono, una condizione di non completa tutela. Si fa riferimento a difficoltà di alcuni testimoni ed imprenditori a mantenere rapporti con il mondo bancario e finanziario, a situazioni patrimoniali e a rapporti societari che, nonostante la *status* di protezione e gli anni trascorsi, non sono stati definiti. E potrei continuare. Signor Sottosegretario, non c'è nessun allarme, bensì un atteggiamento serio e documentato proprio da parte dello Stato,

legge, «misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quella esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio». Sottosegretario, non bisogna riportare delle cifre, ma ricordare chi era Masciari prima: un imprenditore capace, valente, ricco, che aveva una capacità produttiva elevatissima e quindi un tenore di vita elevatissimo; una moglie dentista brava, capace, competente, affermatissima e quindi con un tenore di vita altrettanto elevato. Rimandare a una cifra e renderla pubblica può impressionare,

ad una sicurezza da garantire, Presidente, solo quando da una località protetta ci si trasferisce presso un tribunale per compiere il proprio dovere di testimone di giustizia. La legge fa riferimento globalmente al testimone di giustizia, in qualunque parte del Paese egli si sposti. Confido, Sottosegretario, nella sua attenta valutazione e nella sua buona fede affinché accerti lei tutte le volte che Masciari ha comunicato

alla criminalità organizzata, in uno Stato di diritto, debba essere patrimonio comune e quindi non debba avere alcun colore politico.

hanno dato particolare attenzione e interesse alla ricerca spaziale nazionale, specialmente quella finalizzata allo sviluppo dei sistemi satellitari di comunicazioni cosiddetti a banda larga, consentendo all'Italia di essere di essere completamente presente, con grande rispetto e prestigio, nella ristretta cerchia dei primissimi Paesi «spaziali» del mondo. È doveroso ricordare alcuni tra i più importanti successi italiani nel settore delle comunicazioni via satellite, molti dei quali conseguiti con largo anticipo e con prestazioni non certo meno efficaci rispetto ai corrispondenti prodotti prodotti degli Stati Uniti d'America: il satellite «Sirio 1» nel 1977, preoperativo nelle bande 12-18 i satelliti «Italsat 1» e «Italsat 2» della metà degli anni Ottanta e della metà degli anni Novanta, che hanno sperimentato - primi nel mondo - l'utilizzo della banda larga K e le tecniche digitali di *processing* a bordo dei dati di comunicazione; la piattaforma satellitare multiservizio Artemis, nella seconda metà degli anni Novanta, che ha effettuato sperimentazioni di comunicazioni a banda larga e con grandi volumi di dati, tra diversi satelliti in orbita e la Terra, comprese le prime sperimentazioni di comunicazioni satellitari in mobilità; il sistema di comunicazioni della sonda spaziale «Cassini», che ha rappresentato un mirabile esempio delle eccellenti capacità tecnologiche ed applicative dell'industria italiana. Si può, in questa sede, confermare che il settore delle comunicazioni satellitari a larga banda è, in effetti, una delle aree di maggiore attenzione che il commissario dell'ASI, di recente nomina, è stato chiamato ad analizzare al fine di sottoporre una proposta complessiva di attuazione, sia per quanto attiene gli sviluppi che possono essere sostenuti con fondi nazionali, sia per quanto attiene gli sviluppi che possono derivare da collaborazioni internazionali. Vale a questo riguardo precisare, in via anticipata, che, come primo passo, questo Ministero intende accelerare la realizzazione dell'importante programma satellitare ATHENA-FIDUS (che riguarda essenzialmente lo sviluppo di un satellite di comunicazioni a larga banda, per servizi governativi ed istituzionali, tra cui la telemedicina, la mitigazione del fenomeno sociale del *digital divide*, l'*e*-*government* ed i servizi di infocomunicazioni per la pubblica amministrazione), basato sulla collaborazione istituzionale italo-francese, che coinvolge, anche finanziariamente, i Ministeri della difesa e della ricerca dei due Paesi. Parallelamente, sempre nel settore delle comunicazioni satellitari a larga banda, sarà data priorità agli sviluppi tecnologici e applicativi affinché anche le infrastrutture di terra del sistema ATHENA-FIDUS siano predisposte in tempo per consentire, appena il satellite sarà in orbita, un suo tempestivo utilizzo da parte degli utenti. In tal senso, in collaborazione con il Dipartimento di protezione civile e la Difesa civile, sarà accelerato, e possibilmente ampliato, un primo progetto applicativo per la realizzazione di una rete integrata (terrestre e satellitare)

potrebbe essere estesa a livello europeo per favorire lo sviluppo delle applicazioni governative del programma di navigazione satellitare Galileo e di quello di osservazione della Terra GMES In conclusione, questo Ministero è pienamente consapevole dell'importanza e delle ricadute di questo settore, conferma l'attuazione degli impegni assunti e non mancherà di riferire,

ufficialmente fino adesso, a noi sembra che l'Italia non sia ufficialmente presente nel privato e che gli ultimi spazi venduti siano quelli che, passati da STET a Telecom, quindi a Tronchetti Provera, siano poi passati alla Lehman Brothers di cui oggi si parla molto non in modo particolarmente positivo. Non so se siano poi altri i riferimenti italiani, magari non immediatamente riconoscibili, ma un'attenzione del nostro Governo ad investimenti seri in questo campo così importante per la comunicazione

all'articolo 1, comma 605, ha previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni scolastici 2007-2009; la stessa legge, tuttavia, ne ha subordinato la concreta fattibilità ad una verifica annuale, da condurre d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, in relazione alle compatibilità finanziarie. La legge n. 296 citata ha peraltro previsto una serie di misure atte a realizzare un più razionale utilizzo delle risorse e una maggiore efficienza del sistema dell'istruzione, che avrebbero comportato, nel biennio 2007-2008, un contenimento degli organici di complessive 47.000 unità tra personale docente e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Verificata l'impossibilità di conseguire queste riduzioni in soli due anni,

con la previsione di una riduzione complessiva di posti, tra personale docente ed ATA, di 14.000 unità per l'anno 2007-2008 e di 11.000 unità per ciascuno dei tre anni successivi. Per l'anno scolastico 2008-2009 la medesima legge finanziaria per il 2008 ha disposto un ulteriore contenimento nella misura di 2.000 posti, portando in tal modo a 13.000 unità l'intervento riduttivo da attuare nello stesso anno scolastico, ed ha mantenuto la clausola di salvaguardia che prevede la riduzione delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero, ad eccezione delle competenze spettanti al personale, in misura corrispondente alla quota di riduzioni non operata in ciascun anno. Le riduzioni da operare nell'anno scolastico 2008-2009 sono state suddivise in 12.000 posti per il personale docente e 1.000 per il personale ATA. Non si può quindi prescindere dai vincoli posti dalla legge nonché dalla situazione della pubblica finanza. Di questa situazione si è fatto carico il Governo predisponendo le misure in materia di organizzazione scolastica contenute nell'articolo 64

Il citato articolo 64 prevede, in particolare, l'adozione di un piano programmatico di interventi, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché l'adozione di uno o più regolamenti per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Soltanto a conclusione del percorso delineato dal suddetto articolo 64 potrà dunque farsi una fondata valutazione sul fabbisogno di risorse umane e sulle reali capacità di assorbimento da parte del sistema scolastico, al fine di evitare situazioni di soprannumero e il riprodursi del precariato. Ciò premesso, considerati gli impegni precedentemente presi e la loro sostenibilità in rapporto all'attuale situazione economica e finanziaria del Paese, per il corrente anno scolastico 2008-2009 sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato di 25.000 unità di personale docente ed educativo e di 7.000 unità di personale ATA. Queste assunzioni consentono di corrispondere alle necessità del sistema scolastico salvaguardando, comunque, la qualità del servizio d'istruzione in termini di efficienza ed efficacia. Ricordo infine che le economie di spesa che saranno realizzate in attuazione delle misure previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 saranno destinate, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale del personale della scuola.

che dava all'istruzione un ruolo portante, assegnare solo qualche ora di facciata all'educazione civica, per garantire un po' tutti. Rispetto al quadro europeo, siamo molto colpiti dal fatto che, mentre la Gran Bretagna arriva ad innalzare l'obbligo scolastico a 17 anni, noi ci allontaniamo allontaniamo dagli obiettivi di Lisbona ed abbassiamo l'obbligo a 14 anni, trovandoci quindi in una posizione assolutamente inaccettabile.

al tema degli organici, è certo che, se si taglia ovunque, il primo taglio riguarda proprio gli organici, tra l'altro in modo anche surrettizio: sembra infatti che, dal momento che non si riassumono precari, i tagli non ci siano, come se queste persone fossero anime morte, ma non siamo ai tempi di Gogol.

molto precisi, a volte anche molto difficili; lo ringrazio anche perché in Commissione ha sempre dichiarato quello che pensava, a differenza del Ministro, invece quasi silente.

che mandiamo a casa oltre 200.000 precari. Tra l'altro - mi dispiace anche dirlo - non c'è stata una sola parola sul precariato storico, quello cioè che da dieci anni lavora regolarmente nelle nostre scuole, diploma i nostri figli e rende regolare lo svolgimento delle lezioni,

quando una giovane precaria chiese risposte ai problemi dell'occupazione, lui rispose: «Io, da padre, le consiglio di cercare di sposare il figlio di Berlusconi o un milionario». Questa è l'ultima spiaggia delle giovani insegnanti precarie? E dei giovani insegnanti precari maschi chi si preoccupa? Ineluttabilmente accompagnati a mature ereditiere in sovrappeso, come ci racconta da sempre la letteratura della blasonata commedia all'italiana? Una commedia, appunto, la beffa delle beffe. Tanti, troppi lavoratori obbligati dal precariato all'uscita dal mercato del lavoro via decreto: un biglietto di sola andata per la disperazione. Come si fa, come dice il *Premier*, a reagire con *humour*, quando non puoi permetterti il sorriso di un lavoro e la serenità di un salario? Ma si sa, questo Governo è a favore delle famiglie, della scuola, dell'università e delle donne, quelle donne che ha deciso di mandare a casa perché devono occuparsi dei propri figli, dei figli che stanno in casa perché manca il tempo prolungato, e devono purtroppo essere mandate a casa perché - come si sa

l'atto di sindacato ispettivo in discussione fa riferimento allo schema di decreto inviato dal Ministero agli uffici scolastici regionali con la circolare n. 19 del 1° febbraio 2008, riguardante le disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2008-2009. In particolare, per quanto concerne le dotazioni organiche previste per la Basilicata, l'onorevole senatore interrogante lamenta che le riduzioni operate, rispetto al precedente anno, non terrebbero adeguatamente conto delle caratteristiche geomorfologiche e delle condizioni socio-economiche di quella Regione. Va premesso che il decreto in argomento si è perfezionato con la firma del Ministro dell'economia e delle finanze, oltre che del titolare di questo Dicastero. Esso reca la data del 24 aprile 2008, è stato registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008 ed è stato poi pubblicato nella *Gazzetta* *Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008. Nello stesso decreto è precisato che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che ha rimodulato gli obiettivi di contenimento stabiliti dalla legge finanziaria per il 2007 ed ha previsto per l'anno scolastico 2008-2009 una riduzione complessiva come ho già detto rispondendo alla precedente interrogazione - di 11.000 posti (10.000 per il personale docente e 1.000 per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario). La riduzione incremento di posti relativi al personale docente è stata definita, per ogni Regione, tenendo conto prioritariamente della previsione dell'incremento o del decremento degli alunni e di tutte le altre nuove disposizioni di razionalizzazione previste dalla legge finanziaria 2008. Sono state applicate tutte le misure individuate dalla stessa legge finanziaria per il raggiungimento dell'obiettivo, quali l'innalzamento del rapporto alunni-classe, la riduzione dei posti di docenti specialisti di lingua inglese nella scuola primaria, la possibilità di derogare ai parametri stabiliti per la formazione delle classi; ciò, al fine di evitare l'applicazione della clausola di salvaguardia. Le consequenziali riduzioni di dotazione organica sono state apportate - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - in parte in organico di diritto, per una quota pari al 60 per cento, e la restante quota del 40 per cento in organico di fatto; ciò, per non arrecare grave pregiudizio alla qualità del servizio scolastico e per rispondere meglio alle esigenze del territorio, nonché per avere una maggiore disponibilità di posti utili per la mobilità e per le nomine in ruolo al fine di una maggiore stabilità del personale interessato, a tutela della continuità didattica. Quanto all'esigenza di intese interistituzionali in materia, ricordo che nella suddetta circolare ministeriale n. 19 del 2008 è stata, tra l'altro, segnalata l'opportunità di porre le basi per realizzare intese tra gli uffici scolastici regionali e le Regioni, utili a sviluppare, per l'anno scolastico 2009-2010, una programmazione dell'offerta formativa coerente con l'obiettivo di migliorare sia la qualità del servizio d'istruzione che l'efficienza e l'efficacia della stessa. Da quasi un decennio, infatti, la rete scolastica è rimasta pressoché immutata nelle sue strutture, cioè nei punti di erogazione del servizio e nei centri di coordinamento e di gestione, favorendo così sprechi di risorse, sperequazioni sperequazioni e disfunzioni che occorre superare per rendere pienamente efficienti i servizi scolastici e per raggiungere risultati qualitativi migliori e di più alto profilo. È questo uno degli obiettivi che si prefigge di realizzare lo schema di piano programmatico elaborato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 Tornando alle riduzioni di organico previste nel suddetto decreto interministeriale del 24 aprile 2008, le stesse sono state successivamente verificate sulla base dei dati consolidati relativi al numero degli alunni comunicati dalle scuole tramite il Sistema informativo. All'esito di questa verifica, con nota ministeriale del 4 giugno 2008, è stata comunicata agli uffici scolastici regionali la quota di riduzioni da effettuare in organico di fatto e, successivamente, con circolare n. 58 del 20 giugno 2008, sono state impartite istruzioni ed indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Nella conseguente ripartizione si è tenuto conto dell'andamento delle iscrizioni, che per alcune Regioni ha fatto registrare un minor calo rispetto a quello inizialmente previsto - è il caso della Basilicata - e per altre un minore incremento di alunni rispetto alla previsione utilizzata per la determinazione dell'organico di diritto. Per ciò che si riferisce alla dotazione di posti per le attività di sostegno agli alunni diversamente abili, la legge n. 244 del 2007 - comma 413 dell'articolo 2 stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, il numero massimo dei posti di sostegno, sia in organico di diritto che di fatto, non può superare il 25 per cento del numero complessivo delle sezioni e classi delle scuole attivate nell'anno scolastico 2006-2007. La medesima norma stabilisce, altresì, che per il conseguimento di questo obiettivo vengano definiti criteri e modalità con riguardo alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli allievi disabili anche attraverso compensazioni tra Province diverse e in modo da non superare il rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. Inoltre, al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, il comma 414 del medesimo articolo 2 abolisce la possibilità, prevista dalla legge n. 449 del 1997, che vengano attribuiti posti in deroga al numero di posti assegnato a ciascuna Regione. Le disposizioni contenute nel decreto 24 aprile 2008 tendono dunque a realizzare, anche per quel che concerne le dotazioni organiche per il sostegno, il graduale raggiungimento degli obiettivi previsti dalla suddetta legge. Sulla base del contingente assegnato, ciascun ufficio scolastico regionale ha assicurato la distribuzione degli insegnanti di sostegno in relazione all'effettiva presenza di alunni disabili, tenendo conto anche delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali. Per realizzare pienamente la funzionalità e l'attività delle scuole, gli uffici scolastici regionali - ivi compreso quello della Basilicata - hanno attivato incontri con le Regioni e gli Enti locali al fine di assumere scelte il più possibile condivise in materia di adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuole, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico ed assicurare un più razionale utilizzo delle risorse. Tutto ciò premesso in via generale, per quanto riguarda specificamente la Basilicata faccio presente che la riduzione indicata nella tabella G allegata al decreto del 24 aprile 2008 è stata determinata in base alle suddette disposizioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008 e tenendo conto della diminuzione del numero degli alunni prevista in sede di determinazione dell'organico di diritto. A seguito della verifica del numero degli alunni iscritti alle scuole della Basilicata, effettuata in sede di determinazione dell'organico di fatto per il corrente anno scolastico, tenuto anche conto di quanto rappresentato dall'ufficio scolastico regionale circa le difficoltà logistiche e strutturali esistenti nel territorio regionale, il numero dei posti da ridimensionare in organico di fatto è stato ridotto di 50 unità, come risulta dalla tabella G trasmessa dal Ministero in allegato alla nota protocollo n. 9242 del 4 giugno 2008. Questo per quel che concerne la dotazione organica di personale docente. Per quel che riguarda poi la riorganizzazione generale del sistema scolastico lucano, la direzione scolastica regionale ha riferito di avere più volte indicato all'ente Regione la relativa necessità. Infine, per ciò che concerne il «processo di interazione» in Basilicata tra il sistema di istruzione e quello della formazione, comunico che nell'anno scolastico e formativo 2007-2008 nella stessa Regione sono stati attivati i seguenti percorsi di istruzione e formazione professionale: sei a Potenza e tre a Matera al terzo anno del primo ciclo, a Potenza e quattro a Matera al secondo anno del secondo ciclo, per un totale complessivo di 362 allievi.

la mia piena soddisfazione ed il mio ringraziamento al sottosegretario Pizza per la risposta che ha fornito in relazione all'interrogazione in oggetto. Vorrei ricordare, per dovere di verità, come ha fatto giustamente il sottosegretario Pizza, che il precedente Governo aveva predisposto un taglio che riduceva di 578 posti l'organico dei docenti nella Regione Basilicata, tanto che lo stesso Presidente della Regione, nel febbraio 2008, aveva definito il taglio improvvisato, perché non corredato dall'indicatore di riparto che dovrebbe tener conto dell'entità prevista della popolazione scolastica, nonché del grado di densità demografica, delle condizioni socio-economiche e delle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Il decreto interministeriale del precedente Governo non teneva assolutamente conto dei dati della popolazione scolastica in possesso della Regione Basilicata. assolutamente necessario che si avviasse una riorganizzazione del servizio scolastico in Basilicata, con un'azione concertata tra i vari livelli istituzionali, in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza con la funzione sociale che la scuola ha soprattutto nelle piccole ed isolate comunità del nostro territorio regionale. Quindi, la riduzione di un numero così elevato di posti (578) era stata già predisposta dal precedente Governo. I tagli da loro previsti erano sicuramente maggiori di quelli previsti dall'attuale Governo, come giustamente ha con precisione dichiarato il sottosegretario Pizza. L'azione essenziale di questo Governo mira soprattutto ad assicurare una riqualificazione dell'offerta formativa, con la realizzazione di un sistema educativo in grado di creare i raccordi giusti tra le esigenze del territorio e le politiche nazionali ed europee, nonché la qualificazione della spesa e l'efficienza dei servizi, come ha ben dichiarato il sottosegretario Pizza. La strategia del Governo è quella che qualunque persona di buonsenso farebbe propria: eliminare progressivamente gli sprechi premiando i migliori. La scuola e l'università in generale devono essere luogo di cultura e di formazione. Se oggi funzionano male, o non funzionano affatto, dobbiamo essere consapevoli che per i prossimi decenni avremo una classe dirigente figlia di tali situazioni. In un mondo globalizzato come il nostro, l'unico termine di paragone è rappresentato dalle scuole straniere; è soprattutto con queste che deve avvenire il confronto, non con le nostre "parrocchiette", dove, alla fine, i concorsi li vincono sempre i figli di alcuni padri. Riteniamo quindi che il nostro Governo stia procedendo alla costruzione di un sistema dell'istruzione e della formazione largamente condiviso dalla società civile e dalle rappresentanze sociali e sindacali; quali

riguardanti notizie apprese dalla stampa su alcune tipologie di diplomi di laurea rilasciati dal Politecnico di Torino, si risponde sulla base di elementi informativi riferiti dal rettore. Nelle scelte operative del suddetto Politecnico, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi rappresenta un valore strategico ed è stato quindi ritenuto fondamentale offrire agli studenti italiani la possibilità di una preparazione che possa costituire un vantaggio competitivo sia nell'ottica del proseguimento degli studi, che in quella lavorativa, grazie all'approfondimento della lingua inglese, considerata veicolare soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche. L'ateneo, pertanto,

tutti i corsi di 1° livello che si svolgono presso la sede torinese prevedono, limitatamente al primo anno, la possibilità di optare per una frequenza a lezioni tenute in italiano o in inglese, evitando naturalmente la duplicazioni dei corsi; dal secondo anno i medesimi sono erogati in italiano. Al fine di incentivare gli studenti italiani alla scelta del percorso in lingua inglese, è prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse,

In proposito, si ritiene che tale esonero dal pagamento delle tasse rientri nell'ambito di una autonoma valutazione dell'ateneo, purché il conseguente minor gettito delle entrate non vada a ricadere sull'importo maggiorato della tassazione per gli altri studenti, nonché sulla qualità ed entità dei servizi per i quali sono previsti contributi, come indicato all'articolo 2, comma 2, del citato La mancata previsione del pagamento, ed insieme la sollecitazione verso la scelta di percorsi in lingua inglese, hanno motivazioni di elevato valore formativo e sociale, riferite a specifici *input* del sistema socio-economico e ad un forte interesse del sistema territoriale, anche nell'ottica di una facilitazione nel dialogo con altre realtà universitarie ed imprenditoriali e nell'approccio verso la produzione scientifica internazionale, dove la lingua inglese è quella maggiormente adottata. Pertanto, l'agevolazione economica riconosciuta non può qualificarsi come una discriminazione verso gli altri studenti italiani proprio perché, in funzione del suo obiettivo, rappresenta un incentivo per quegli studenti che si propongono per percorsi formativi più impegnativi e non determina conseguenze negative a livello professionale per l'inserimento nel mercato del lavoro italiano ma, al contrario, favorisce l'inserimento medesimo nel mercato globalizzato. Nei confronti degli studenti stranieri che seguono corsi in inglese, il piano di studi prevede, comunque, che la loro formazione tecnica sia completata da quella linguistica in italiano con lo specifico obbligo, nel percorso di studi, del superamento di un insegnamento di lingua e cultura italiana, al quale è attribuito il valore di dieci crediti. Non esiste, in realtà, alcun danno per la lingua e la cultura italiana come conseguenza delle azioni poste in essere dall'ateneo, che al fine di perseguire i suoi obiettivi istituzionali mira ad una formazione dei propri studenti tale che in futuro possano operare al meglio quale classe dirigente di un mondo internazionalizzato: nel mondo reale di oggi, infatti, la marginalizzazione è data proprio dalla difficoltà di interfacciarsi, anche a livello linguistico, con il resto del mondo. La conferma di quanto esposto si rileva dalle richieste che provengono dal mondo del lavoro, aziende nazionali ed internazionali, di personale laureato con conoscenze linguistiche di carattere professionale. Riguardo il corpo docente si precisa che, pur non essendo di madrelingua inglese, è professionalmente preparato per la realizzazione dei percorsi formativi in parola. Si ritiene, pertanto, che scelte diverse da parte del Politecnico di Torino, risulterebbero anacronistiche e che, quindi, le opportunità offerte agli studenti, anche riguardo alla formazione in lingua inglese, siano assolutamente positive per il loro futuro, com'è d'altronde dimostrato dalla crescita del tasso di iscrizione a fronte del calo demografico. Per una più completa informazione sull'organizzazione dei corsi in parola, si riferisce quanto segue: i corsi di laurea di 1° livello in ingegneria dell'autoveicolo si svolgono sia in italiano che in inglese; il corso di laurea in ingegneria tessile presso la sede di Biella è svolto in inglese; tale scelta è dovuta a specifici *input* del sistema socioeconomico anche da ascrivere ad una rispondenza più qualificante della preparazione alle richieste di mercato. Per i corsi di primo livello presso la sede di Vercelli viene proposto un primo anno sia in italiano che in inglese; dal secondo i corsi di laurea in ingegneria civile e meccanica si svolgono in italiano, mentre quelli in ingegneria elettronica in inglese.

*(PD)*. Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per essersi fatto portavoce del rettore perché mi pare che, più che aver avuto un'impressione o un giudizio del Governo, abbiamo appreso

quindi, a capire quale sia la posizione del Governo italiano relativamente a questa decisione che, per come è stata riassunta nella nella risposta data, sembra andare nella direzione di formazione di personale altamente qualificato e specializzato perché vi è una domanda di un determinato tipo di specializzazione. Non si prende in considerazione il fatto che

essere, visto e considerato che in questo Paese - ahinoi! - esiste il valore legale dei titoli di studio, la necessità di portare a casa un pezzo di carta. Come però non siano saltati agli occhi gli elementi di discriminazione nei confronti di chi

mi pare preoccupante. Questo, tra l'altro, è un Governo che ha fatto dell'italianità non soltanto una bandiera della campagna elettorale, ma anche un motivo per il quale alcune delle nostre imprese non avrebbero mai dovuto cadere nelle mani degli stranieri. In questo caso, però, non si prende in considerazione il percorso umano, culturale, ma anche economico di chi arriva a 19 anni conoscendo bene una lingua e di chi, invece, arriva a 19 anni non conoscendo bene una lingua. È molto più probabile che qualcuno abbia appreso la lingua recandosi all'estero piuttosto che studiandola in Italia; è molto più probabile che chi ha la possibilità di recarsi all'estero abbia uno

Quindi, se qualcuno oggi in Piemonte volesse studiare ingegneria tessile lo può fare soltanto nella lingua di Shakespeare. Io non ho assolutamente niente contro la lingua di Shakespeare essendomi laureato in letteratura nordamericana e parlando altre tre o quattro lingue, ma questo non mi deve far avere un accesso privilegiato a un servizio scolastico scolastico pubblico. Torneremo sulla questione perché, oltre a tutto ciò che abbiamo cercato di evidenziare nella nostra interrogazione relativamente alla discriminazione nei confronti di chi non ha potuto, per vari motivi che non devono interessare lo Stato, studiare una lingua, ci sono degli aspetti economici della disuguaglianza linguistica - di cui noi italiani già soffriamo, vista la qualità dell'insegnamento delle lingue in Italia

dei concetti che non appartengono alla nostra cultura. Sempre con l'associazione esperantista radicale stiamo preparando una proposta di legge di tutela e promozione della lingua italiana. Io le ho portato uno studio

l'insegnamento delle lingue. Tra i 27 Stati membri ce ne é uno, la Gran Bretagna, che ne porta a casa un'ampia fetta. Se veramente abbiamo a cuore il sistema educativo italiano, e anche l'italianità, perché tra opera tra opera lirica e opere di letteratura l'Italia non ha sicuramente niente da invidiare a nessuno, forse bisognerà prendere in considerazione anche l'aspetto della lingua italiana, oltre a tutto ciò che le ruota intorno.

Grazie